la norma proposta al comma 1 dell'articolo 11 del decreto che stiamo discutendo sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale verrà applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, che passerebbe così dal 21 al 22 per cento. Il termine attuale era stato fissato lo scorso luglio al 1° luglio 2013. Con un debito pubblico da *record* (secondo Eurostat, nel primo trimestre del 2013 il rapporto debito-PIL ha raggiunto nel nostro Paese quota 130,3 per cento, e ci vede superati solo dalla Grecia in questa non certo invidiabile classifica), il provvedimento sull'IVA, pur con un evidente moto di prudenza, appare inevitabile se non si vuole infliggere una mazzata definitiva ai consumi che, vorrei ricordare, sono pari all'80 per cento del PIL (fonte Confcommercio), senza naturalmente dimenticare che un eventuale aumento dell'IVA colpirebbe soprattutto e in particolare le fasce più deboli e gli incapienti. Del resto, sappiamo tutti molto bene che con l'attuale livello di pressione fiscale ogni possibilità di crescita economica del nostro Paese è seriamente compromessa, se non inesistente. Di fronte ad una recessione che colpisce tutti i settori produttivi del Paese, la strada della riduzione fiscale deve essere obbligata essere obbligata e dovrà necessariamente passare attraverso una seria riforma del sistema fiscale che approdi ad una semplificazione e alla riduzione del costo degli adempimenti. Il rinvio dell'aumento dell'IVA lascerebbe, per il momento, più soldi in tasca agli italiani, consentendoci di rispettare i vincoli di bilancio, ma come ha tenuto a precisare il portavoce del commissario agli affari economici Olli Rehn, la Commissione UE ha bisogno di capire «come coprire il buco nei conti che si crea con il rinvio dell'IVA prima di commentare la misura». Sarà quindi necessario, e inevitabile, capire come coprire quel buco, magari cercando una soluzione che vada oltre ogni rinvio e che permetta di trovare le risorse per cancellare definitivamente l'aumento dell'IVA. Ci si può provare pensando ad una revisione specifica e mirata della *spending review* o ad un'accelerazione della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare; una *spending review* che non sia solo un annuncio, come è avvenuto con il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, che in pratica ha proceduto solo a dei tagli lineari della spesa. La revisione della spesa è un'operazione straordinaria e come tale va affrontata, investendo tempo (almeno un anno, dicono gli esperti) e investendo risorse per pagare dei professionisti che devono elaborare una sorta di piano strategico per ciascun settore e che devono avere un forte sostegno politico. Probabilmente negli anni 2011 e 2012 l'emergenza in cui si è trovato il nostro Paese ha impedito questa operazione ma credo sia arrivato il momento di investire risorse e capitale politico. Non possiamo più permetterci di attendere; soprattutto, basta frasi ad effetto e sparate giornaliere, che vanno rimandate con coraggio al mittente, in particolare se questo è il nostro alleato politico. Per l'anno in corso è prevista un'ulteriore contrazione dei consumi del 3 per cento, insieme ad un aumento della povertà assoluta. Di fronte a questo quadro, i segnali di ripresa per il 2013 sono davvero difficili da vedere. allora avere il coraggio di progettare e non solo di gestire; bisogna avere il coraggio dì dire che il problema degli italiani non è l'IMU sulla prima casa, perché gli studi ci dicono il contrario. Bisogna magari avere il coraggio dì prendere anche decisioni impopolari, ma che vadano nella direzione giusta, che riducano la forbice della disuguaglianza che rende i ricchi sempre più ricchi e ì poveri sempre più poveri. Diceva ieri un collega del Movimento 5 Stelle che abbiamo ridotto di 7,6 milioni il Fondo per il funzionamento ordinario delle università; di fatto, non vengono ridotti gli stanziamenti alle università, ma vengono aumentati, in quanto per la stessa cifra finanziamo, all'articolo 2, le attività di tirocinio durante il corso degli studi di laurea per rendere effettiva l'alternanza tra studio e lavoro. Lo stanziamento previsto è di 3 milioni per il 2013 e 7,6 milioni per il 2014. Quindi, con questo decreto si prevede un aumento di risorse per le università e non un taglio. Una collega della Lega ieri affermava che con questo decreto foraggiamo di nuovo le Regioni poco virtuose, come la Campania; ciò non corrisponde al vero, perché i commi 13 e 16 dell'articolo 11 integrano le disposizioni per la procedura di accertamento dei disavanzi e, di conseguenza, la definizione dei piani di rientro in materia di trasporto ferroviario regionale della Regione Campania. I piani di rientro si realizzeranno in cinque anni e hanno come finalità la riorganizzazione e la riqualificazione del sistema di mobilità regionale su ferro. Le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Concludo con quanto contenuto nel Manifesto delle giovani classi dirigenti: occorre procedere a un ricambio generazionale delle classi dirigenti del Paese per fare in modo che la ripresa economica parta dal potenziale dei giovani; il Paese, per innovare e modernizzare, deve necessariamente attingere a quello che possiamo definire il potenziale inespresso dei suoi trenta-quarantenni.

nostro esame contiene misure importanti, e particolarmente importante è un elemento richiesto dal Popolo della Libertà, ma certamente condiviso, anzi l'annullamento dell'aumento dell'IVA: un aumento che probabilmente non avrebbe portato maggiore gettito perché avrebbe causato una diminuzione dei nostri consumi, per cui avrebbe semplicemente contribuito a deprimerli, con tutto a deprimerli, con tutto quello che ne consegue anche a livello di mero gettito per lo Stato, senza creare beneficio. Pertanto, meritoriamente, l'IVA non aumenterà. Il provvedimento contiene anche norme per la promozione dell'occupazione,

il Governo Monti pensò di ricavare del denaro, necessario a migliorare i saldi del nostro bilancio, aumentando a dismisura

di questa imposizione, di 150 milioni di euro; naturalmente tutto ciò doveva andare a bilanciare delle spese e così via. La realtà è che, anziché incassare 150 milioni, se ne incassarono 13; il il danno però fu molto superiore a quei 137 milioni di euro mancanti. Non erano previsioni sbagliate nel senso che si era valutata male la platea,

vuol dire che oltre il 90 per cento delle imbarcazioni da diporto sono state o rottamate o spostate all'estero; pertanto, anziché creare un beneficio di 13 milioni per lo Stato (non è quello il beneficio), si è creato un grave danno, perché tutto l'indotto, tutte le spese che sono connesse

viene introdotta una specifica tassazione sulle sigarette elettroniche. Spero che il Sottosegretario, impegnato nelle carte, riesca anche ad ascoltarmi; non dubito delle sue capacità e a lei mi rivolgo in quanto rappresentante del Governo. È sicuro il Governo che stabilendo questa imposizione il gettito aumenterà e non diminuirà invece? Ho constatato con stupore che nessuno ha pensato di consultare, anzi neppure di avere dei dati attendibili su quale sia oggi in Italia il mercato delle sigarette elettroniche. Quando

rilevante *export*, ha affermato che una tassazione di questo genere, non solo per l'entità ma più ancora per le modalità con le quali viene introdotta, causerà probabilmente la chiusura di migliaia di negozi, dunque la perdita di migliaia di posti di lavoro, e anche la cessazione dell'attività di molti impianti che producono queste sostanze. impianti lavorano anche per l'esportazione, ma nel momento in cui il mercato italiano sarà desertificato, poiché - com'è noto - la tassazione, il costo del lavoro, le condizioni generali non sono particolarmente favorevoli in Italia rispetto agli altri Paesi

migliaia di posti di lavoro, gettito per lo Stato in termini di imposta sul reddito e finiremo per perdere anche

(perché dovranno essere sottoposte allo stesso regime di coloro che vendono tabacchi e sigarette ordinarie), verosimilmente migliaia di questi negozi chiuderanno,

Nel momento in cui rimanesse questo rifiuto, coloro che lo esprimono se ne assumono la responsabilità: se fra un anno queste migliaia di posti di lavoro saranno persi, bisognerà che qualcuno venga a spiegare perché ha detto no a queste proposte e ha «ucciso» migliaia di posti di lavoro.

ovvero relativamente alla copertura finanziaria degli interventi, parere favorevole con osservazioni. L'esame degli oltre 700 emendamenti predisposti a più riprese è stato impegnativo e si ringrazia il personale dell'Ufficio, che ha sopportato me, in quanto relatrice, e gli altri Commissari in modo puntuale e preciso. La legge che stiamo approvando contiene numerosi interventi di variegata natura, ma il pacchetto più rilevante riguarda gli interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile. puntano ad incentivare i datori di lavoro ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ad incentivare il contratto di apprendistato professionale ed a promuovere tirocini formativi. misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, il Piano di azione coesione, disposizioni in materia di istruzione e formazione e quant'altro in materia di rapporti di lavoro. L'attuazione di tutte queste misure porterà ad un incremento netto della base occupazionale giovanile e ad una maggiore qualificazione delle potenzialità lavorative. Voglio qui soffermarmi solo su uno di questi settori di intervento, ovvero sulle disposizioni sui tirocini formativi, e fare una raccomandazione al Governo sull'inserimento della dimensione di genere nei provvedimenti che riguardano il mondo del lavoro. Per quanto riguarda i tirocini formativi,

e alle amministrazioni un'iniezione di entusiasmo e innovazione, anche se qualche volta sono stati utilizzati in modo improprio per sostituire personale vacante.

anche per l'Università è previsto un incentivo sulla base di un accordo specifico (3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 per il 2014). L'unica nota dolente riguarda le altre amministrazioni pubbliche, che agli oneri derivanti da questa misura devono provvedere utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio, attingendo prioritariamente ai fondi destinati al finanziamento di incarichi e consulenze, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Questo è un problema: occorre segnalare che l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che la spesa per incarichi e consulenze debba essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella registrata a consuntivo nell'esercizio 2009. Si tratta pertanto di capitoli di spesa ben poco ulteriormente comprimibili; pertanto, se si vuole davvero incentivare il tirocini a livello locale occorre trovare un'altra modalità di copertura. Vengo alla raccomandazione al Governo di inserire la dimensione di genere all'interno dei provvedimenti riguardanti il lavoro. La lettura del tasso di occupazione, di disoccupazione e del numero di giovani che smettono di cercare un lavoro fornisce una base informativa dalla quale partire per delineare le politiche, che risulta molto più chiara se letta con la dimensione di genere. Le giovani donne hanno tassi di occupazione più bassi, tassi di disoccupazione più alti e, soprattutto al Sud, rinunciano maggiormente a cercare un lavoro, che è il vero sintomo della sfiducia nei confronti del mondo del lavoro ma anche del riconoscimento dei propri talenti. Nella difficile situazione che stiamo vivendo, anziché avvicinarci ci stiamo allontanando dall'Obiettivo di Lisbona del 60 per cento di occupazione femminile. In alcune zone d'Italia, in particolare le zone urbane del Nord, la percentuale di donne occupate si avvicina all'obiettivo, mentre al Sud il divario si fa più drammatico. Abbiamo tutti insieme firmato la Convenzione di Istanbul e parliamo ogni giorno di contrasto alla violenza alle donne: ebbene, il miglior modo di contrastare gli abusi in famiglia è quello di dare dignità alle donne attraverso il lavoro e l'indipendenza economica, che consente loro di sottrarsi alle situazioni di violenza. Tuttavia, non voglio qui assumere la difesa di una categoria svantaggiata, bensì far notare che il lavoro delle donne è un vantaggio per l'intera collettività. Tutti gli studi dimostrano che un aumento consistente del PIL passa attraverso l'incremento del lavoro delle donne; che tutte le organizzazioni risentono positivamente di un *mix* equilibrato tra i generi; che la creazione di un posto di lavoro femminile ha un effetto moltiplicatore di 1,3, perché una donna che lavora ha bisogno di aiuto in casa, se ha figli necessita di una *baby-sitter*, acquista cibi pronti e altro ancora. In conclusione, chiedo al Governo una maggiore attenzione alla dimensione di genere,

se vogliamo anche in modo schizofrenico, gli stessi interventi che sono ormai presenti nella letteratura in materia di politica del lavoro da alcuni decenni. di interventi che si sono resi utili a tratti, prevalentemente per sostenere un'economia in crescita e per brevi periodi,

In modo particolare, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del

anzi, diciamo di più, l'incentivazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, come nel caso dell'articolo 1,

Signor Presidente, il brusìo accompagna quest'Aula sempre. Qualche volta sarebbe anche utile capire perché un decreto-legge, che quindi è già legge, individui la categoria dei giovani che vivono soli con una o più persone a carico; carico; a leggerlo in italiano sembrerebbe un assurdo: come fa un giovane a vivere solo e avere anche una o più persone a carico?

Parliamo di occupazione aggiuntiva in ragione di un netto che è frutto di una media degli ultimi 12 mesi, fatte salve le diminuzioni anche delle società controllate o partecipate del soggetto che ha assunto.

Magari è anche giusto. Magari siamo costretti a fare così perché siamo tutti europei, siamo tutti a favore del libero mercato, ma ci fa comodo utilizzare la leva del denaro pubblico per aiutare le nostre imprese. Magari è giusto,

rapporti di lavoro stabili ma, al tempo stesso, favoriamo molto, non poco, la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro perché le imprese utilizzino quello strumento. E badate, facciamo qualcosa di veramente insopportabile. Sapete cosa sono i tirocini formativi e di orientamento? Sono strumenti nati per consentire un'esperienza di lavoro volontaria ai giovani nell'interesse dei giovani, e sono stabiliti dei parametri per cui a fianco al giovane che viene preparato deve essere presente un *tutor*; non c'è soggetto pubblico o privato che non abbia da rispettare un rapporto tra tirocinanti e lavoratori a tempo indeterminato e con esperienza all'interno dell'azienda. noi trasformiamo il tirocinio formativo e di orientamento, Ministro, in una brutta fattispecie, in una modalità di sfruttamento

una umidità di illegalità che viene legalizzata dalle leggi, che anche noi contribuiamo a varare e che non risolvono il problema: lo lasciano lì e, in aggiunta, introducono elementi culturali negativi. Dopo che tutti quanti noi ci siamo spesi per sostenere che bisogna qualificare i giovani per dare loro una prospettiva,

a giovani non in possesso di diploma di scuola media superiore e neanche di scuola professionale. Noi dobbiamo spendere di più e meglio i nostri soldi, anche privandoci di qualche privilegio che pure abbiamo accumulato, per investirli in favore dei giovani e togliere

È un provvedimento manifesto che noi speriamo il Governo voglia cambiare.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo un lungo e tortuoso *iter*, svolto anche e soprattutto in Commissione, giunge oggi in quest'Aula il provvedimento a tutti noto come «decreto sul rinvio dell'IVA». Il testo, in realtà, si divide in due importanti sezioni che trattano di altrettanti rilevanti ed importanti temi: il lavoro, con alcune disposizioni che puntualmente ed inesorabilmente finiscono a svantaggio del Nord, e, per l'appunto, il rinvio sull'IVA. Su uno dei due punti, il lavoro, ad eccezione dell'intervento sulla riforma Fornero (riforma che tutti hanno subito), per cancellarne gli effetti negativi sui contratti a termine, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, non crediamo si possano condividere le altre misure adottate per rilanciare l'occupazione, per il semplice motivo che la strategia perseguita da questo Governo in materia di politiche per l'impiego continua a caratterizzarsi di assistenzialismo per il Sud, sottraendo quindi risorse al Nord. risorse stanziate e gli incentivi previsti, infatti, finiscono per sussidiare soltanto giovani meridionali che non hanno proseguito gli studi e ai quali non diamo, quindi, nemmeno possibilità di crescita o di studio successivo e che non vivono più con la famiglia d'origine.

Non più tardi di un mese fa, infatti, colleghi, il Ministro dello sviluppo economico, nel corso dell'assemblea di una importante associazione di categoria, affermò che gli sarebbe piaciuto evitarlo, ma non c'era scelta: l'IVA sarebbe aumentata di un punto a partire da luglio. Vibranti furono allora le contestazioni di chi era presente in sala, soprattutto perché solo chi lavora, cercando con fatica di salvarsi da questa crisi devastante, sa benissimo che cosa comporterebbe un aumento percentuale dell'aliquota ordinaria dell'IVA: l'ennesimo ed inevitabile crollo dei consumi! Sì, perché questo Governo, a partire dal Ministro dello sviluppo economico, farebbe bene a leggersi i risultati consolidati del gettito delle imposte indirette dei primi cinque mesi del

l'IVA che in un anno ha permesso allo Stato, proprio per l'alto livello di questa imposta, di non incassare quasi 3 miliardi di euro, una cifra importante per il Paese in questo momento di crisi notevole. Un ammanco incredibile causato - guarda caso - da una flessione della domanda interna. I cittadini, insomma, a causa dell'alta tassazione e alle poche entrate dovute ad una serie di motivi che credo siano a voi noti, non consumano, ovvero non comprano, e non comprando il gettito dell'imposta diminuisce e gli imprenditori, i piccoli artigiani, i commercianti, chiudono l'attività. Ecco perché, onorevoli colleghi, quel giorno i presenti in sala hanno protestato: perché più aumentano le tasse, più aumenta l'IVA, più le aziende muoiono. E più le aziende cessano, più aumenterà la disoccupazione, ovvero quel dramma del lavoro che contate di che contate di risolvere con le disposizioni contenute all'interno di questo stesso provvedimento: il più classico esempio del cane che si morde la coda! Non si può quindi essere soddisfatti della decisione assunta dall'Esecutivo all'interno di questo provvedimento, perché la buona notizia del rinvio da luglio ad ottobre dell'aumento dell'IVA non risolve il problema, ma lo sposta solo in avanti di qualche settimana. Continua a regnare, insomma, l'incertezza, la regola che questo Governo ha ormai assunto, ovvero il non scegliere. Un'incertezza che si accompagna, peraltro, anche ad una iniquità. Come per il precedente Esecutivo, infatti, anche per questo Governo le tasse sono come le ciliegie: una tira l'altra. E così, l'unica copertura finanziaria trovata per sospendere l'IVA quale è stata? L'aumento degli anticipi di IRPEF ed IRAP. Ma che grande idea, che grande novità, che capacità di salvare questo Paese! Forse potevamo pensarci prima o forse era meglio evitare questo tipo di intervento - e mi rivolgo al Governo - con azioni che sono ancora più vessatorie nei confronti di aziende che devono dare lavoro. Quando e come possono dare lavoro, se stanno chiudendo? Non aumentare l'IVA, temendo un ulteriore crollo dei consumi da parte dei contribuenti, per aumentare gli anticipi di tassazione su contribuenti ed aziende: della serie, con una mano vi diamo qualcosa, con l'altra vi prendiamo il doppio!

anche per questo provvedimento il Governo cosa ha scelto? Il rinvio, l'ennesima non scelta. Questo valzer di posticipi e sospensioni, tuttavia, è ormai arrivato al termine, onorevoli colleghi. Siamo arrivati a fine luglio

nelle varie Regioni): la Sicilia, un territorio ricco di mare, di sole e con un patrimonio architettonico di inestimabile valore distribuito in un'area di circa 26.000 Un territorio spesso offeso, maltrattato, il cui patrimonio culturale è frutto di un contatto con popoli assai diversi, un contatto spesso poco armonioso. In Sicilia sono arrivati i Sicani, i Siculi, i Greci, i Romani, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Svevi, i Francesi e gli Spagnoli. È una terra piena di riserve naturali. Ne elenco solo qualcuna: l'Isola Bella di Taormina, la riserva naturale del Monte Pellegrino, la riserva dello Zingaro,

Faccio anche un breve sunto delle bellezze architettoniche, dei monumenti più importanti. Perché non pensare ai templi di Agrigento, di Segesta, di Selinunte, splendidi mosaici della villa del Casale di Piazza Armerina? Perché non ricordare poi i superbi duomi di Palermo, di Cefalù, di Monreale, il barocco siciliano, che non è solo quello della Val di Noto, la cittadina punica di Erice, Mozia? E non continuiamo, ci fermiamo solo a questo. Chiedo a lei, signor Presidente (lo faccio in maniera virtuale, perché so che non possiamo aprire una discussione in questo momento), e a tutti voi senatori, cari colleghi distratti di quest'Aula: è possibile che in questo Paese non si possa vivere di turismo? del giorno di oggi reca: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare quella giovanile

Sto dicendo tutta una serie di cose semplici, non rivoluzionarie, e intanto ancora non ne parliamo. Insisto: con la *green economy* e l'industria blu si possono trovare migliaia di posti di lavoro per i giovani nei servizi turistici, nella tutela del territorio, nei beni artistici, nel mercato agroalimentare e dell'artigianato, divenendo un'occasione formidabile di formazione e di primo impiego per l'Italia, per l'Italia intera. Lo scorso Governo tecnico ha fatto stringere la cinghia a tutti, lo ha fatto davvero; tanto è vero che persone semplici, cittadini semplici come me hanno deciso di venire qui per cercare di cambiare o di dare una mano a voi che siete esperti nel cambiare

sono state esautorate dai decreti-legge arrivati la sera per l'indomani, impedendo alle persone semplici e normali come noi di capire qual era il sistema per poter modificare e contribuire fattivamente a migliorare quest'Italia. sono bloccate da altro atteggiamento. L'ostruzionismo vero, signor Presidente, non è il nostro, ma quello che il Governo e questa maggioranza stanno mettendo in atto:

intanto loro li hanno ritirati, non pensando agli interessi degli italiani e dei cittadini, non pensando che ancora oggi la gente muore per questo sviluppo insostenibile e non tollerabile

È iscritta a parlare la senatrice Mussolini. Ne ha facoltà.

propri delle Commissioni permanenti, proprio per dare risposte ed esaminare questo testo che parla di occupazione giovanile e di lavoro stabile. Esso consente ai datori di lavoro di ottenere incentivi per giovani dai 18 ai 29 anni

con un lavoro a tempo determinato. In questo caso si offre loro non solo un'occasione di lavoro, ma anche stabilità e tranquillità sociale.

perché dicono che non c'è una prospettiva di crescita. Allora, diamo fiducia a questi provvedimenti, aperti come maggioranza - ma ho visto anche come Governo, da parte dei Ministri e degli stessi Sottosegretari - a ulteriori miglioramenti.

che contengono nicotina o altri succedanei, e che assolutamente non si debba introdurre questa tassazione estremamente pesante (il 58,5

aumento di consumo, ma sempre se non viene aumentata la tassazione su questo prodotto, che certamente sta andando bene. Ci sono tanti produttori, molti negozi,

molti degli interventi che mi hanno preceduto hanno ribadito che il termine «giovani» in larghe parti del nostro Paese non rappresenta più da tempo quell'età lavorativa che arriva fino ai 24-25 anni, ma neppure ai 29. Si sposta invece sempre più oltre i 35 e i 40, a quella che dovrebbe essere invece l'età di piena affermazione professionale delle persone. Quando parliamo di giovani, in particolare nel Mezzogiorno, parliamo quindi di fasce anagrafiche tra loro diverse. È un punto, questo, che non può essere sottovalutato, e restare fermi all'interno della fascia dei 29 anni, come il decreto-legge oggi in esame è quasi costretto a fare per un ordine di priorità dei problemi, ma anche per il necessario riferimento a norme comunitarie, non cogliere appieno l'ansia di quei trentenni per i quali diventa sempre più difficile inserirsi nel mondo del lavoro senza incentivi economici. Ecco perché io credo che, almeno per i percorsi di alta formazione, è necessario e si può, già oggi nella conversione del decreto-legge, del decreto-legge, portare la soglia di incentivo fino almeno ai 32 anni. Tra l'altro, l'età media dei nostri laureati a conclusione della specialistica è di 27 anni per i maschi e di 26 anni per le donne. Questi sono soltanto dati di media. Mi sembra avanzi pochissimo tempo per stare dentro i 29 anni che danno la possibilità degli incentivi. Il decreto‑legge oggi in esame fa una scelta promuovendo l'occupazione stabile dei giovani, specialmente di quelli che si trovano in particolari situazioni di svantaggio. svantaggio. Ancora una volta, però, dobbiamo constatare l'esiguità delle risorse, indubbiamente neppure lontanamente sufficienti a superare uno dei problemi più pesanti del nostro Paese. Eppure, è da apprezzare che le scelte che il Governo propone vanno nel senso da noi auspicato di impegnare maggiori risorse, almeno tra quelle disponibili, per il Mezzogiorno e per i soggetti svantaggiati.

Sarebbe come se, siccome le risorse oggi a disposizione possono aiutare solo alcune decine di migliaia di persone, a fronte delle centinaia di migliaia di giovani che ne avrebbero bisogno, ai primi

Diciamo quindi: scarse risorse sì, ma strumenti importanti, in particolare se accompagnati da risorse aggiuntive, e forse importanti soprattutto per il futuro.

su tutto il territorio nazionale, anche se sull'apprendistato dobbiamo dire che per ridare tale ruolo a questo contratto occorre, salvo rare eccezioni, depotenziare in prospettiva tutte quelle forme contrattuali, magari meno vincolanti e meno costose, ma che difficilmente possono dare al giovane la speranza di un percorso professionale stabile. Mi avvio rapidamente alle conclusioni, con due motivi di riflessione. Il primo riguarda l'abrogazione dell'aliquota agevolata al 4 per cento delle cooperative sociali e dei loro consorzi, come previsto dalla legge di stabilità per il 2013. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, con la cooperazione sociale parliamo di un pezzo fondamentale di *welfare* del nostro Paese. L'aumento dell'IVA al 10 per cento, operante dal 1° gennaio del prossimo anno, rischia di compromettere la stessa esistenza di molte cooperative sociali, con la perdita di lavoro di molti lavoratori e la cessazione di importanti servizi sociali sul territorio. Se il provvedimento che andremo a votare oggi non potrà contenere l'abrogazione del comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità, mi auguro che che almeno possa esserci l'impegno del Governo a tornare sul tema con la legge di stabilità per il 2014, senza chiusure anticipate, ovviamente, ma anche senza pregiudizi. Passo al secondo e ultimo motivo di riflessione: in tema di lavoro giovanile, credo che occorra ragionare sulla crisi ma anche sul futuro e sulle prospettive future degli attuali giovani.

zii e nonni, di essere messi nella condizione di avere un giorno una pensione equa e dignitosa, cosa complicata con un percorso professionale a singhiozzo, precario, con più o meno lunghi periodi di disoccupazione. Per questo motivo, tra l'altro, occorre rivedere per esempio i costi di recupero a fini contributivi della laurea, da troppi anni diventati proibitivi per la maggioranza dei lavoratori. Non si è coerenti con il richiamo all'impegno agli studi per i più giovani, se poi non si permette di far valere quell'impegno anche a fini contributivi. Anche per questa ragione, non è un caso che la laurea possa essere considerata da troppi giovani come un inutile appesantimento di vita, un ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, un'ulteriore perdita di anni di contribuzione.

relativamente al fondo ordinario. Pertanto, quell'elemento di polemica mi sembra poco significativo.

nel nostro Paese purtroppo ci sono molti laureati e molte persone con alta specializzazione disoccupati da più di sei mesi, che non hanno un lavoro regolarmente retribuito da più di sei mesi. Quindi, non c'è un'esclusione di questo tipo.

per dare ai giovani di questo Paese, in una situazione di grave crisi, che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi

Dovremo affrontare la questione degli esodati, ma anche quella relativa alle piccole mobilità. Pensate cosa significa per le aziende sotto i 15 dipendenti non disporre più dello strumento che permetteva a questi lavoratori di avere un incentivo per la rioccupabilità.

sulle cosiddette sigarette elettroniche potrebbe tra l'altro comportare il problema di incentivare il ritorno all'utilizzo della sigaretta normale. Questo, a mio avviso, e secondo quanto segnalato dalla relazione della Commissione sanità, potrebbe comportare un non indifferente problema per il sistema sanitario e per la disincentivazione del tabagismo, con eventuali possibili costi di tutto rispetto. In secondo ho udito le proteste più che vibrate per l'aumento degli acconti per le imprese e per le persone fisiche. Mi sembra opportuno qui ribadire - e non certo *ad adiuvandum* della disposizione - quanto già sinteticamente segnalato nella mia relazione, e cioè il contribuente può comunque determinare l'acconto in via presuntiva. Ad esempio,

vi è stata una sensibile diminuzione degli affari, che comporterà un'imposta di soli 100 euro, tale sarà l'entità del suo acconto; se addirittura va in negativo, il contribuente Da ultimo, desidero ringraziare non solo tutti gli intervenuti, ma anche e soprattutto i componenti delle Commissioni, che si sono fatti non solo in quattro per questo provvedimento, ma addirittura in otto. Signor Presidente, ho un'istanza da rivolgere. Le chiedo cortesemente di sospendere la seduta

dalla fine degli anni Novanta si registra un preoccupante calo delle popolazioni di api, bombi e altri insetti impollinatori in tutti i continenti, con picchi di sconcertante gravità del fenomeno in Europa e Nord America. Com'è noto, le api rivestono un ruolo chiave nel ciclo della vita, essendo alla base del delicato processo di impollinazione delle piante. Infatti, in assenza delle api o nel caso di una loro drastica riduzione numerica la produzione di cibo su scala globale subirebbe una consistente flessione, con conseguenze drammatiche, sia per gli esseri umani che per gli animali. I seguenti dati devono essere presi in considerazione: fino al 35 per cento della produzione di cibo a livello globale dipende dal servizio di impollinazione naturale offerto da questi insetti; delle 100 colture da cui dipende il 90 per cento della produzione mondiale di cibo, 71 sono legate al lavoro di impollinazione delle api; solo in Europa, ben 4.000 diverse colture dipendono dall'impollinazione entomofila; per cento delle 264 specie coltivate in Europa sono frutto dell'impollinazione naturale operata da api, bombi, farfalle e falene; i benefici economici a livello globale legati all'impollinazione naturale ammontano a circa 256 miliardi di euro. Il declino delle api è attribuito a diversi fattori, tra cui l'uso agricolo di neonicotinoidi, che costituiscono una classe di insetticidi sistemici di nuova concezione che negli ultimi 15 anni ha conosciuto una rapida diffusione. Studi come quello del progetto APENT e il rapporto pubblicato, il 16 gennaio 2013, dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, condannano i rischi che i pesticidi neonicotinoidi comportano per le api e, in particolare, accertano il danno provocato da tre di queste sostanze (clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam). Quanto detto conferma quello che apicoltori, cittadini e associazioni denunciano da anni. Numerosi apicoltori testimoniano che, una volta interrotto l'uso di tali sostanze, le api ricominciano naturalmente a ripopolare i campi. I neonicotinoidi, in ragione del loro elevato rischio di neurotossicità, oltre a rappresentare una minaccia per insetti utili come le api, potrebbero rappresentare anche un possibile rischio per la salute dei vertebrati, compreso l'uomo. Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli studi che vedono nei neonicotinoidi una potenziale fonte di alterazioni sottili anche sui vertebrati, rischio che dovrebbe essere adeguatamente valutato con particolare riguardo agli effetti neuroendocrini. L'Istituto superiore di sanità di Roma già nel 2009 sottolineava che gli effetti neuroendocrini dei neonicotinoidi nei vertebrati meritano una più attenta valutazione in relazione ai potenziali rischi. In linea generale, soggetti particolarmente vulnerabili come bambini, donne in gravidanza, soggetti con alterazioni endocrino-metaboliche, risulterebbero maggiormente esposti attraverso la diffusione di questi principi attivi nell'ambiente, nelle filiere alimentari e, quindi, anche nei prodotti dell'alveare. Per i soggetti adulti, infine, è documentata l'azione inibente dei neurotossici sulla capacità riproduttiva e sulla fertilità maschile umane. Inoltre, la caratterizzazione dei possibili rischi per la salute umana associati all'esposizione a interferenti endocrini è attualmente definita una una delle nuove priorità per la sicurezza degli alimenti e dell'ambiente dall'Istituto superiore di sanità. Ciò premesso, appare evidente come il tentativo, ad opera di multinazionali operanti nel settore dei pesticidi, di attribuire il declino delle api a svariate cause patologiche specifiche apistiche si possa spiegare alla luce dell'intento di proteggere gli enormi proventi economici derivanti dalla vendita di tali prodotti, a scapito della sopravvivenza di una specie animale di incommensurabile valore per il genere umano. In particolare, i pesticidi più pericolosi sono sette: si tratta di neonicotinoidi e altre sostanze i cui brevetti sono di proprietà di colossi chimici come Bayer, Syngenta, BASF e altre ancora. In Italia, il Ministero della salute ha prorogato, con decreto del 25 gennaio 2013, fino al 30 giugno 2013, la sospensione dell'autorizzazione d'uso dei concianti sistemici sul mais. Sebbene il divieto in questione abbia dato immediatamente un respiro di sollievo alla popolazione di api, la proroga di tale sospensione è ormai scaduta e il problema si ripresenta in tutta la sua gravità. A livello europeo, il recente regolamento n. 485 del 2013 istituisce restrizioni all'utilizzo di tre neonicotinoidi per limitarne l'impatto negativo sulle api. Tuttavia, le relative restrizioni si applicheranno solo dal 1° dicembre 2013 e, ad ogni modo, il provvedimento ha carattere transitorio, arrivando a coprire un periodo di due anni. In sintesi, l'uso di questi insetticidi è l'unico fattore di totale responsabilità umana su cui un intervento legislativo possa produrre effetti diretti e verificabili. Bisogna agire in fretta per evitare che nel periodo di agosto-dicembre 2013, in assenza di uno specifico divieto di utilizzo di tali prodotti, venga inferto un altro duro colpo al patrimonio apistico nazionale. In ragione della gravità della situazione e delle potenziali conseguenze, è necessario trovare una soluzione definitiva al problema, mirando ad impedire in maniera permanente l'utilizzo l'utilizzo di prodotti con le citate componenti chimiche nel nostro Paese. A questo scopo ho depositato un'interrogazione urgente al Ministro della salute e al Ministro delle politiche agricole e forestali.

ci sentiamo delegittimati nelle nostre funzioni di parlamentari e soprattutto ci sentiamo indignati come rappresentanti dei cittadini e rappresentanti di questo Stato.